Comunico che, in data 4 dicembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rassegnate dall'on. Galeazzo BIGNAMI.

pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1272, di conversione in legge del decreto-legge 17 recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, è convertito in legge con le modificazioni riportate

Signor Presidente, questo decreto nasce con delle intenzioni del tutto condivisibili, perché sburocratizzare è sempre cosa buona e il settore dell'ambiente sta vivendo delle sfide tali per cui è sicuramente necessario aggiustare la normativa e migliorarla in funzione di quello che ci riserva il futuro. i contenuti di questo decreto e il modo in cui è stato esposto confermano drammaticamente che questa maggioranza avanza per mantra, e cioè continua a ripetere ossessivamente delle cose che servono sostanzialmente per catturare l'attenzione del suo elettorato. Qui il mantra fondamentale usato è quello di essere contro il *green*: è un decreto sull'ambiente, ma bisogna essere contro il *green*, anche se poi di fatto si approvano delle norme che ovviamente conciliano la conservazione ambientale con le attività umane. È proprio questo il punto e l'ha detto bene ieri la senatrice Minasi nel suo peraltro irreprensibile intervento: le norme *green* erano state approvate in una certa epoca, ma poi sono sopraggiunte altre esigenze di cui adesso bisogna tenere conto. Le norme *green* nascono già

è chiaro che poi nel tempo c'è la necessità di riaggiustarle e di migliorarle, ma non per questo bisogna rinnegarle, perché le norme *green* sono il fondamento del nostro futuro. Essere contro è soltanto utile per catturare l'attenzione di determinate persone deviando però il discorso di fondo, cioè la mentalità che dovrebbe esserci in tutti noi di sviluppare una una cultura di conservazione ambientale. Questo mantra è probabilmente secondo solo a quello che viene continuamente ripetuto, per cui ci si domanda in passato cosa abbiano fatto i Governi della sinistra. Ma io vorrei in questa occasione ribadire il fatto che dal 1992, ovvero da Tangentopoli in poi, la destra ha governato molto di più della sinistra, per cui ci sarebbe da chiedersi cosa è successo quando governava la destra. *(Applausi)*. Questo lo dico perché non lo dice mai nessuno e qualcuno prima o poi deve anche dirlo. Un altro punto che secondo me è discutibilissimo nel decreto in esame è quello dell'accentramento del potere nel Ministero e nel Governo. Si continua a parlare sempre - come si è fatto anche in altri casi in passato - dei commissari governativi che vengono nominati con i pieni poteri e che scendono dall'alto, in del loro cavallo bianco, e aggiustano tutto. Ebbene, non funziona esattamente così e questa volontà di affermazione del centralismo statale con la volontà manifestata sempre da questa maggioranza di sviluppare le autonomie: o si va verso le autonomie o si va verso l'accentramento. Io rappresento un territorio, l'Alto Adige, che ha una sua competenza in alcuni settori molto legati all'ambiente, come la Protezione civile. Per cortesia, non mandateci commissari governativi, ce la caviamo benissimo da soli. questo dimostra che ci sono competenze che sarebbe meglio lasciare alle Regioni, anziché accentrarle nel Ministero. Nel decreto-legge in esame, invece, le Regioni vengono usate esclusivamente per eseguire gli ordini che arrivano dal centro e poi, se non funzionano, per essere riprese, soprattutto se sono amministrate da governi di un colore diverso rispetto al Governo romano. Inoltre vengono usate come raccoglitori di dati, perché dopo il Ministero li rielabora con la sua grande saggezza. Io credo che questa grande saggezza centralista non porti a molto. Ripeto ancora una volta che è necessario rafforzare le autonomie decisionali locali nel settore della tutela dell'ambiente, per sviluppare quella cultura di cui dicevo prima, che sicuramente non si crea continuando a parlare soltanto di commissari governativi.

rispetto alla fase preindustriale; il livello del mare si è alzato di 30 centimetri sulla costa degli Stati Uniti; la temperatura media è diversa da zona per zona sulla Terra ed è diverso anche l'innalzamento del livello del mare, ma ci sono zone dove viene misurato in cui l'innalzamento è forte. Si prevede addirittura che l'Oceano Atlantico si alzi di due metri entro il 2100. Ricordiamo che la gran parte della popolazione vive sulle coste. Pertanto tutto questo inciderà sulla presenza umana sulle coste. Per non parlare poi del fatto che il riscaldamento globale - qualcuno non ci pensa - vale quanto migliaia di bombe atomiche fatte precipitare sui nostri oceani. Ciò comporta il riscaldamento di grandi masse d'acqua, che poi si scontrano con altre grandi masse d'acqua fredda e si formano gli uragani; pertanto, dal riscaldamento globale nascono gli uragani.

quella città, e invase il territorio interno, che era agricolo, sommergendo la strada storica che collegava Grado ad Aquileia

tutta la parte meridionale del Lazio, creando una grande palude. Mi sembra che non sarebbe una cosa buona, ma soprattutto che si dovrebbero creare i presupposti per poter affrontare situazioni emergenziali di questo tipo.

Mi sembra che questi aspetti andrebbero considerati, e invece non si fa nulla. Il PD ha proposto la costituzione di zone di interesse strategico per poter fare impianti anche di grandi dimensioni, per ovviare a questo: penso, ad esempio, ai desalinizzatori, perché l'acqua c'è, è nel mare e ce ne sarà sempre di più; per poterla utilizzare in agricoltura bisogna desalinizzarla. Ma questo evidentemente non si può fare se non si costruiscono grandi impianti, e già mi prefiguro le discussioni pubbliche quando si deciderà di farne, perché sarà necessario e non si potrà più rinviare.

voi avete scelto una certa strada. Noi abbiamo presentato degli emendamenti perché avremmo voluto interloquire su quella strada. Voi avete deciso che le autorizzazioni saranno soltanto dei grandi impianti che producono energia,

gli impianti che sono stati autorizzati e su cui abbiamo fatto dei modesti passi in avanti sono piccoli e molti legati al superbonus. Poi decidete di cambiare completamente strategia,

vi siete accorti che nel frattempo avete fatto altri decreti? Il decreto ambiente cozza in maniera irreversibile - tanto che io vedo il blocco e neanche l'autorizzazione degli impianti grandi - con il decreto agricoltura

il provvedimento originario per normare la materia dell'energia - dite esattamente l'opposto. Gli *stakeholder* che in questi mesi hanno presentato i progetti a chi devono credere? A quelli che stabiliscono, di fatto, che il piccolo è bello, oppure a questo che dice che il piccolo non verrà più neanche valutato e si va direttamente ai grandi impianti?

di altri provvedimenti, ci veniva detto: alt, ci sarà un decreto che si occuperà solo di questo. Ve ne siete però occupati in maniera marginale, anche su temi fondamentali. uno su tutti, quello delle terre rare. È vero che c'è una norma, ma gli stessi soggetti che in Italia fanno del riciclo delle terre rare la loro professione principale sono abbastanza delusi da quell'articolo.

Non mi sembra che Ursula von der Leyen in questi anni abbia fatto delle critiche al Green new deal; anzi, l'ha rappresentato tale e quale alla sua platea, che lo ha votato, anche quello che fu, perché l'appena nominato vice presidente Fitto sarà costretto ad assecondare questa visione. Ma, se si vogliono fare delle modifiche, si deve anche tener conto che in questo Paese ci sono delle eccellenze straordinarie sull'economia circolare, ci sono delle *start-up* innovative per quanto riguarda la *green economy*, che ogni anno riempiono la Fiera di Rimini - lei lo sa benissimo, Vice Ministro - e che rendono il nostro Paese all'avanguardia nel mondo e che meriterebbero un po' più di rispetto. È vero che c'è un'industria tradizionale che merita di essere salvaguardata e deve essere vista con con altrettanta lungimiranza. In questo decreto non c'è nulla sull'industria tradizionale e come portarla a una transizione ecologica, per cui stamattina stanno manifestando i lavoratori dell'Ansaldo e quelli di Leonardo, che chiedono dei rinnovi contrattuali seri, un adeguamento dello stipendio, e sono anche preoccupati per la loro industria e quei lavoratori vanno rispettati.

Infine, vorrei tornare su un emendamento che è stato ritirato - lo dico ai colleghi della Camera, visto che secondo il ministro Ciriani verrà rivalutato e secondo il relatore Rosso verrà addirittura presentato nella legge di bilancio - che è il 3.22, a prima firma del senatore Paroli, sull'affidamento *in house* dei servizi idrici. Lo dico innanzitutto perché ho apprezzato la raffinatezza del Ministro che ha detto che verrà rivalutato. Il collega e amico Roberto Rosso sa che, da quando è stata approvata la riforma della legge di bilancio, le norme di carattere generale non possono essere presentate, ma vengono presentati soltanto articoli ed emendamenti che riguardano il bilancio dello Stato, per l'appunto, e quindi ci sarà un altro provvedimento non meglio definito. Ma anche se si rivalutasse in questo provvedimento non meglio definito, io sommessamente consiglierei al ministro Pichetto Fratin e a questa maggioranza di studiare bene la materia. Capisco Capisco che ci sono emergenze locali che probabilmente hanno determinato questo emendamento; alcuni parlano della situazione presente a Vercelli, e io penso anche un po' alla Sicilia, ma a pensar male si fa peccato ovviamente. Il tema è che oggi l'affidamento *in house* del sistema idrico è molto più complicato, perché il PNRR riguarda anche il sistema idrico e uno può anche dire che il privato non gestisce. Ma che cosa mi rappresenta che il privato non gestisce? Se c'è il privato, c'è il privato e, visto

(quindi anche in forma di SpA, ma il soggetto è pubblico), il PNRR è l'unica cosa che in questo momento fa sbloccare i cantieri nel nostro Paese. Per cui voi potete raccontare in televisione che gli occupati in Italia sono aumentati. se togliete anche quelle risorse, andrete nei programmi televisivi a dire che forse potevate aumentare gli occupati, ma avete preferito risolvere il problema della Sicilia e di Vercelli, per cui avete bloccato tutto. Fate soltanto attenzione, perché su un tema così delicato si creerebbe un precedente per cui un privato viene avvantaggiato rispetto ad altri e temo che gli altri non la prenderebbero bene. Visto che un ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, o una procedura di infrazione con una notifica direttamente all'Unione europea non si nega mai a nessuno, rischieremmo di veder così sfumata la possibilità di investire in questo Paese. Mi spiace per il voto di fiducia, perché di fatto non c'è stata approvazione di nostri emendamenti: si vede che non siamo stati all'altezza di questo provvedimento, anche se devo dire che un po' tutte le opposizioni sono state bastonate ed anche alla maggioranza non è andata meglio. Quindi il nostro voto, anche solo per solidarietà Grazie

colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, sono due anni che chiediamo al Governo di agire sull'emergenza climatica e implementare un vero cambio di paradigma, un nuovo approccio rispetto al cambiamento climatico in atto. due anni chiediamo di mettere in cima alla propria agenda politica tutte quelle urgenti e necessarie azioni di adattamento e mitigazione atte

nelle sfide che il mondo reale, fuori da quest'Aula, ci chiede da tempo di affrontare con competenza. Dopo più di due anni e oltre 70 decreti-legge che normalmente andrebbero emanati eccezionalmente e adottati solo in casi di straordinaria necessità, dopo una miriade di provvedimenti inutili che non sto qui a elencare, arriva in Assemblea anche il decreto-legge sulla tutela ambientale. Sarebbe quasi un sogno poter dire che finalmente si interviene su un'emergenza in atto. Invece, purtroppo no. Questo decreto-legge in perfetto stile *greenwashing* utilizza la parola ambiente come una maschera per nascondere un grave arretramento in materia di politiche climatiche e di transizione energetica. una vera presa in giro e intanto che ci fate perdere tempo andando a peggiorare il presente e il futuro nostro e delle giovani generazioni il Paese rimane in balia delle vere emergenze, quali quali il dissesto idrogeologico e la crisi climatica, che in una sorta di miraggio speravamo di leggere in qualche modo nel provvedimento Purtroppo, colleghe e colleghi, sappiamo bene che questo decreto-legge non solo rappresenta un attacco alla transizione ecologica, ma stringe anche l'Italia ancora di più nella morsa tossica della dipendenza dai combustibili fossili. Per voi della maggioranza è tutela ambientale ridurre la distanza di protezione dalle coste per permettere le trivellazioni marine nel Paese che vanta il *record* europeo per la sua eccezionale e preziosissima biodiversità, ma con il 70 per cento di ecosistemi naturali che nel frattempo sono in pericolo per la loro fragilità. La distanza di protezione ora viene ridotta da 12 a 9 miglia dalla costa. Vi ricordate lo sblocca trivelle di due anni fa nel decreto aiuti-*quater*? Per fronteggiare la crisi energetica, colleghe e colleghi della maggioranza, avete consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi fossili tra le 9 e le 12 miglia. Adesso arriviamo a sole 9 miglia dalle coste. Vogliamo vedere dove si arriverà alla fine della legislatura. Avete anche il coraggio di chiamare tutela ambientale l'emissione delle concessioni per gli idrocarburi e gli incentivi per sfruttare giacimenti esistenti, che avete sempre inserito nella disposizione cosiddetta sblocca trivelle del 2022 con l'intenzione di attingere alle poche riserve di idrocarburi, oltretutto - ci risulta - di pessima qualità. Con un emendamento del relatore permetterete anche di vendere il gas stoccato oltre il termine precedentemente fissato del 31 ottobre 2025. Tradotto in parole semplici, sempre per tutelare l'ambiente - secondo voi - continuerete a dare priorità al veleno (cioè alle fonti fossili) per venderlo alla rete, prolungando la dipendenza dal gas e rallentando di fatto la transizione verso le rinnovabili. Complimenti! A questo punto mi sono chiesta e vi chiedo che definizione avete di ambiente e di tutela ambientale. Per questo, per rinfrescarci la memoria, ritengo utile citare la definizione di Treccani: «La tutela dell'ambiente ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell'aria, dell'acqua e del terreno dovuta a inquinamento, radiazioni o altri residui industriali e agricoli; di preservare l'integrità dei processi naturali minacciata dagli effetti dell'industrializzazione, dell'agricoltura, dello sviluppo commerciale e di altre attività dell'uomo». Penso che sia una definizione chiara, a meno che non contestiate anche questa, cari colleghi. In questo decreto-legge, di fatto, tutelate palesemente le *lobby* dei combustibili fossili, a cui il Governo Meloni proprio non riesce a dire di no, in un atteggiamento fatemelo dire - di vera sudditanza e obbedienza, in un decreto, poi, sulla tutela ambientale: un vero ossimoro, un vero insulto all'intelligenza e uno schiaffo a tutti quei comparti agricoli e industriali che stanno vivendo sulla loro pelle la difficoltà e la difficoltà e i costi legati al cambiamento climatico. Praticamente state curando la ferita con il veleno che l'ha causata. Colleghe e colleghi, questo non è progresso: è suicidio climatico, è un insulto agli impegni internazionali che il Governo ha sottoscritto, è un tradimento nei confronti delle generazioni più giovani. Ma vi siete chiesti in che Italia li costringiamo a vivere? Li costringiamo a vivere in un'Italia del paradosso, in cui gli impianti eolici *offshore* vengono ostacolati da vincoli rigidissimi, mentre invece le piattaforme petrolifere possono avvicinarsi sempre di più alle nostre meravigliose coste. Grazie al TAR del Lazio - e grazie veramente al TAR del Lazio - proprio in questi giorni è stato bloccato l'assurdo progetto di trivellazione nelle acque del delta del Po - ve lo avevamo già ricordato due anni fa una riserva di biosfera, un luogo straordinario riconosciuto come patrimonio UNESCO. Il ricorso è stato presentato anche da nove Comuni del Polesano, traditi dallo stesso Stato che li dovrebbe proteggere. Zero scrupoli sul nostro capitale naturale, zero rimorsi in un territorio, il Polesine, che ha già dato tanto. Grazie al TAR questo scempio è stato fermato. Ma francamente, veramente francamente, non se ne può più di continuare a operare in questo modo obsoleto, figlio di una mentalità dei tempi che furono. Invece il Governo insiste e persiste. Sordo ad ogni appello ed evidenza, permette proroghe praticamente illimitate a tutto: alle concessioni di coltivazione di idrocarburi, che - ricordo - sono quelli che contribuiscono di più in assoluto alla crisi climatica non le temutissime auto elettriche, non gli attivisti che volete arrestare con il disegno di legge sicurezza, non le rinnovabili che osteggiate con tutte le vostre forze. Il bello qui è che sapete benissimo che le conseguenze di queste politiche miopi - politiche che seguono la vecchia mentalità del fare come abbiamo sempre fatto, tanto da chiederci cosa state facendo di diverso rispetto al passato - invece di investire in soluzioni innovative, stanno andando ben oltre il problema della crisi climatica, perché colpiscono direttamente la salute e la vita delle persone. Non smetterò mai di ricordarvi in quest'Aula che ogni anno circa 60.000 persone muoiono prematuramente a causa dell'inquinamento atmosferico, delle polveri sottili e del particolato. Sono 140 i morti al giorno, ma sembra che a voi non interessino: una tragedia silenziosa, che evidentemente non suscita l'attenzione di questo Governo. Che importa se la Corte di giustizia europea ha già condannato l'Italia per il superamento sistematico dei limiti di biossido di azoto? Che importa ridurre le emissioni per migliorare la qualità dell'aria e proteggere la salute di cittadine e cittadini? E che importa inoltre il dissesto idrogeologico, una delle emergenze più gravi del nostro Paese? Non ve ne è traccia né menzione, in questo decreto. E allora avanti con la logica del cerotto sulle emergenze e stop ad approcci sistemici, scientifici e lungimiranti. Questo è il motto della maggioranza ormai da due anni. Colleghe e colleghi, noi di AVS non ci arrendiamo: crediamo e sappiamo che ci sono altre strade; che mettano al centro della propria agenda politica la salute delle persone, il futuro delle nuove generazioni, la crisi climatica, il contrasto al dissesto idrogeologico e le innovazioni e che rispettino, per esempio, la volontà popolare sull'acqua pubblica. pubblica. È doveroso anche per me intervenire sull'emendamento di Forza Italia volto a riaprire le porte alla privatizzazione delle società idriche pubbliche, favorendo i profitti privati a scapito di un bene comune essenziale come l'acqua. Colleghe e colleghi, nella prima bozza di questo decreto-legge ambiente avete provato a inserire un attacco all'acqua pubblica: l'avete cancellato nella seconda bozza, per poi farlo presentare - meschinamente, lasciatemelo dire - sotto forma di un emendamento da un unico senatore di Forza Italia. Avete il coraggio di farlo proprio oggi, mentre la crisi climatica rende l'acqua sempre più scarsa e preziosa, mettendo in ginocchio intere regioni. Quello che esce dalla porta rientra dalla finestra e solo grazie al lavoro delle opposizioni vi siete fermati e avete ritirato l'emendamento in questione.

L'acqua è vita e appartiene a tutte e tutti noi e noi di AVS continueremo a batterci per difenderla e a vigilare affinché il Governo e la destra non ci riprovino.

Signor Presidente, ricordato che il decreto-legge in esame ha avuto un ampio riscontro positivo e l'apprezzamento da parte di tutti gli *stakeholders*, che l'intento del provvedimento è accelerare i tempi per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che si è posto il nostro Paese e che la volontà di questa maggioranza è di aumentare la competitività delle nostre imprese,

quell'esperienza fa capire che non si può continuare a lottare con previsioni normative che non aiutano l'agibilità nel risolvere i problemi che si ha la responsabilità di risolvere. Questo è il caso dell'emendamento già evocato, il 3.22, da me presentato, perché la disposizione revocata anche dal Consiglio di Stato dice chiaramente - purtroppo - che, nel settore dei servizi idrici, sino a quando la specifica disposizione di una legge nazionale non stabilirà la possibilità per i privati di partecipare a una società *in house*, indicando anche la misura della partecipazione e la modalità di ingresso del socio privato, nonché il ruolo all'interno della società e i rapporti con il socio pubblico,

È una società privata, perché è quotata in borsa, o è una società che si può occupare, come sta già facendo, a scadenza, del servizio idrico integrato? Noi dobbiamo decidere questo, non gridare «attenzione all'acqua pubblica». L'acqua è e è e rimarrà pubblica, ci mancherebbe che qualcuno lo mettesse in discussione, ma la gestione dev'essere aperta ai privati, altrimenti ci troviamo nella situazione che ci ricorda la Banca mondiale, le dispersioni idriche nelle reti dei Paesi ad alto reddito si aggirano intorno al 10-20 per cento. In Italia il dato è del 40 due quinti dell'acqua immessa nella rete finiscono nel terreno, si disperdono. Il 22 marzo del 2024, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, l'Istituto di statistica ha pubblicato i dati sullo stato della rete idrica, confermando questo *trend*:

Continuiamo così? Mi sono preso la briga di capire perché in Italia ci sia questa dispersione. Tutti gli operatori dicono chiaramente che la responsabilità è del basso livello di investimento e della bassa capacità da parte del pubblico di intervenire. O prendiamo questa notizia come un dato, e ci lavoriamo, oppure continuano a gridare «acqua pubblica, acqua pubblica», ma il risultato è che l'acqua non c'è, perché non arriva. esiste l'amministrazione privata delegata e sono in maggioranza aziende con partecipazione privata. In Francia esiste la gestione privata delegata

le medesime siano partecipate dagli enti locali, che il socio privato, selezionato mediante procedure di evidenza pubblica, detenga, direttamente o indirettamente, una quota del capitale sociale non superiore a un quinto e che non gli spetti l'esercizio di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società. È forse un attacco all'acqua pubblica o è la collaborazione di privati? Che nel 2024, quasi 2025, in Italia si abbia ancora paura del privato è qualcosa che ritengo intollerabile e inspiegabile. Davvero non possiamo pensare di andare in questa direzione ancora per lungo tempo. Il secondo tema che volevo affrontare è un po' più spinoso: è un richiamo che voglio fare alla mia maggioranza,

possiamo accettare che il 3 dicembre su questi emendamenti non ci sia ancora un parere del MEF e ci ritroviamo a non poterli discutere? *(Applausi)*. Con responsabilità li ritiriamo, ma questa cosa non può continuare. Li abbiamo ritirati, perché siamo responsabili, ma, per una comune responsabilità che abbiamo, dobbiamo migliorare questo rapporto tra Governo e Parlamento. Così non si può andare avanti, perché l'unica lettura rischia di diventare una mezza lettura

ci dia la possibilità, il prima possibile, di rimediare alle mancanze, alle dimenticanze e a ciò che non abbiamo affrontato adeguatamente, è chiaro che continueremo ad essere costruttivi e collaborativi, ma nella chiarezza e nella serietà che credo sia scontata per tutti noi. Abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione. Forza Italia si considera comunque soddisfatta e voterà a favore della fiducia, evidentemente. È un provvedimento che abbiamo costruito insieme alla maggioranza,

i relatori, il Presidente della Commissione e chi del Governo si è dato da fare per costruire una positività, che c'è stata, ma purtroppo è stata parziale, rimando ad altre occasioni in cui

anni, ma non abbiamo più tempo. Con questo auspicio, confermando il voto favorevole di Forza Italia, rinnoviamo la nostra disponibilità a costruire insieme soluzioni migliori.

perché volevamo metterci a disposizione per tutte le possibili misure da adottare per la tutela dell'ambiente, la promozione dell'economia circolare e la gestione delle risorse idriche, per le semplificazioni nei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, per le disposizioni di bonifica dei siti contaminati e per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Concetti aulici, signor Presidente, ma privi di grande impatto e, come poi vedremo, vuoti di contenuti.

e gli emendamenti tra l'altro lasciavano intendere che nemmeno il Governo fosse poi tanto a conoscenza di quello che stava succedendo, nonostante li avesse varati in prima persona, è inutile nasconderlo. Ecco che abbiamo assistito al valzer degli emendamenti accantonati,

ricordo che il MoVimento 5 Stelle ha presentato quasi 90 emendamenti, tutti annullati o azzerati, tranne per la magnanima concessione di qualche ordine del giorno,

e ne hanno già parlato anche altri colleghi, ma è un punto fondamentale. Ritengo che l'inefficienza della pubblica amministrazione non debba essere l'alibi per dare ai privati maggiore spazio di manovra. *(Applausi)*. Ricordo che la gestione del pubblico in molti Comuni e in molte Regioni è in mano alle vostre forze politiche, non certo al MoVimento 5 Stelle, quindi mi sembra più un alibi che altro. I cittadini italiani hanno già ha ribadito,

nulla ha messo in campo, ma ha soltanto messo in risalto le difficoltà politiche - le abbiamo sentite - della maggioranza, ma anche strutturali di questo Paese, a cui ancora una volta, però, il Governo non ha saputo porre rimedio. Gli *stakeholder* ci hanno fatto presente, per esempio, che la rete infrastrutturale

elogio i risultati che abbiamo portato a casa attraverso gli emendamenti che sono stati approvati. Il mio intervento sarà coerente e rinnovabile, per usare un termine

poco serio che tiene nei confronti degli elettori e dei cittadini, abbia travisato e interpretato in maniera molto opportunista linee politiche che essa stessa ha condiviso, propalato e propinato come verità assolute. Proprio in queste ore, questo cortocircuito - per rimanere in tema elettrico - sta manifestando tutta la la concretezza delle nostre teorie: proprio poche ore fa la Regione Sardegna ha definito una mappa delle aree idonee all'installazione degli impianti impianti di produzione di energia rinnovabile. Questo è il primo cortocircuito, perché mi sembra che proprio coloro i quali amministrano la Regione Sardegna siano stati quelli che manifestavano con le loro bandiere il sostegno all'atteggiamento inquisitorio portato avanti da manifestazioni internazionaliste come quella di Greta Thunberg, tralasciando aspetti che noi della Lega avevamo anticipato in tempi non sospetti. Penso al tema della sostenibilità di misure che - nessuno lo può negare - stanno indirizzando, anche vincolandolo, il sistema produttivo per il raggiungimento di obiettivi che, nella condominialità europea e anche internazionale, l'Italia ha sottoscritto. Non ho ancora sentito parlare, specialmente da parte delle opposizioni,

la distinzione tra potenza e tensione: non tutto ciò che produce energia consente di ottimizzare, in termini di tensione, la necessità di fornire energia, specie ai settori energivori del sistema produttivo del nostro Paese;

manteniamo la barra su questo tipo di impostazione. Elogio ulteriormente il Governo per aver ricordato che c'è spazio anche per lo sfruttamento della diversificazione delle fonti di approvvigionamento di energia in tema di nucleare. Su questo abbiamo previsto almeno 5 gigawatt nella prima ipotesi e 20 nella seconda, per poter fornire energia programmabile. Qui c'è un altro risultato importante ottenuto in sede di conversione: tra le priorità tra le priorità che potranno essere oggetto di accelerazione in sede di esame VIA-VAS, abbiamo inserito il cosiddetto pompaggio, cioè quel sistema che, grazie agli invasi,

un accenno storico - fu riconosciuta anche dal primo ministro Winston Churchill, che nel 1941 volle addirittura provare a sabotarlo per far mancare l'acqua al Meridione d'Italia. In questo testo

che è stato nominato per tirare fuori l'Italia dalla grande serie di infrazioni che ci sono state comminate dall'Europa sul tema delle acque reflue

Amichevolmente lo voglio soprannominare capitan disgrazia, perché sembra che, secondo la sua lettura, in questo Paese si possano motivare decine di scioperi a settimana,

Non dubito che la CGIL promuoverà subito un altro sciopero di fronte a questi atti concreti del Governo. Non ho sentito parlare neppure del tema della neutralità climatica. Ricordo gli obiettivi del Fit for 55, che ci vedono impegnati - anche qui, volenti o nolenti - al rispetto di determinati obiettivi. Dobbiamo essere attenti a non

dovuto ricredersi in merito all'assoluta autonomia e autosufficienza di tante misure che noi riteniamo invece di dover attentamente osservare. Mi Mi sembra che la coerenza di questo provvedimento si possa assolutamente esprimere con il grande investimento che consentiamo alle

con tutti i settori produttivi, con decine di aziende pubbliche e private, con i cosiddetti *stakeholder* che ci hanno rappresentato moltissime

alla possibilità di dare voce alle tante segnalazioni che abbiamo raccolto e a cui non abbiamo comprensibilmente potuto dare voce, perché ci sono anche i limiti oggettivi del rispetto delle forme nella redazione di decretazione d'urgenza. Non possiamo ovviamente stravolgere i contenuti definiti per ovvie ragioni e quindi siamo impegnati sin d'ora a

Il decreto-legge di cui discutiamo meritava un confronto aperto con le opposizioni, un confronto ampio, serio e approfondito. Sul futuro dell'ambiente ci sarebbe bisogno sempre di equilibrio, responsabilità e condivisione, ma all'Esecutivo questo non interessa. Pure sulle questioni ambientali, infatti, il Governo è un misto di negazionismo, ambiguità, malafede, nostalgia del passato e intolleranza per la sostenibilità. L'articolo 9 della Costituzione, al suo ultimo comma, sancisce che la Repubblica tutela sancisce che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Nonostante questo, il Governo è sordo, rigido e autoreferenziale, e autoreferenziale, non pensa ai giovani e ha un'idea distorta della democrazia e del futuro. Questo Governo osteggia la transizione ecologica ed energetica e noi lo denunciamo con chiarezza. Non solo, rifiutate che l'Italia sia una Repubblica parlamentare, non accettate il bilanciamento dei poteri, vorreste sottomettere la magistratura e la stampa, mirate ad aumentare le disuguaglianze, non volete controlli e agite perché il Capo dello Stato non sia più arbitro istituzionale e garante della Costituzione. Tra l'altro, il Governo Meloni è già nella storia, perché abusa della fiducia parlamentare, nasconde il proprio vuoto interno con parole e frasi *spot*, non sopporta gli impegni sovranazionali e chiunque la pensi diversamente e si muove sempre in maniera confusa e contraddittoria anche nei consessi internazionali. Il *menu* di oggi è un decreto-legge, ribattezzato «ambiente», ma anche questo è pura propaganda e nulla di più. Infatti, il provvedimento ha un contenuto limitato, non affronta le grandi questioni della transizione energetica ed ecologica, né ha l'organicità e la completezza che occorrerebbero per proteggere l'ambiente e raggiungere la neutralità climatica. Questo decreto-legge si occupa di valutazioni ambientali per accelerare i progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che sono già due grandi fallimenti del Governo e della sua maggioranza. Insomma, è un'ennesima toppa in zona Cesarini, per così dire, visti i gravi ritardi accumulati dalla squadra della Presidente del Consiglio. Ancora, questo decreto-legge introduce la definizione di «acque affinate» con l'intento di contribuire a ravvenare le falde, ma senza programmi e risorse per il futuro sul punto. sul punto. Il testo interviene poi sui rifiuti con alcune semplificazioni, ma non sostiene davvero la gestione ambientale. Inoltre, rafforza i poteri, ma non gli strumenti in capo ai Presidenti di Regione riguardo al dissesto idrogeologico. Se non bastasse, il provvedimento vincola fortemente i proponenti di progetti produttivi di energie rinnovabili ed esclude tecnologie innovative: penso ad esempio all'eolico *offshore* o al fotovoltaico galleggiante tra quelle beneficiarie di corsia preferenziale Il decreto-legge, insomma, non appare affatto coerente con gli obiettivi di transizione energetica che l'Italia si è data nel quadro europeo e internazionale. Soprattutto, le norme di questo decreto rischiano di ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, favorendo in maniera indiretta le fonti fossili. Queste criticità erano ampiamente prevedibili, anzi scontate su questo decreto. Infatti, proprio alla recente conferenza sul clima COP29 di Baku, la Presidente del Consiglio dei ministri ha trascurato l'abbandono progressivo delle fonti fossili, già centrate nell'Accordo di Parigi. Inoltre, Meloni ha enfatizzato tecnologie, come il gas fossile e i biocarburanti, marginali rispetto alle rinnovabili, ma soprattutto la presidente del Consiglio ha compiuto una mossa incredibile, parlando di fusione nucleare, dunque sconfessando platealmente il proprio Ministro dell'ambiente e i suoi vice presidenti Salvini e Tajani, fortemente legati alla fissione nucleare. *(Applausi)*. Evidentemente, Meloni ha voluto stupire con effetti speciali, pensando che nessuno si accorgesse della sparata e della contraddizione; così, ha cercato di schermare le idee confuse del Governo rispetto agli sforzi internazionali per la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale. È l'ulteriore conferma della doppiezza di questo Governo, vittima di cortocircuiti interni e diviso pure sulla fusione nucleare, che noi del Partito Democratico siamo stati i primi a sostenere, sapendo che è un investimento e una speranza per il futuro. In questi due anni di legislatura il primo a portare le parole

dite con chiarezza che siete divisi *(Applausi)*, perché c'è un pezzo importante del Governo che parla della fissione nucleare e la Presidente del Consiglio, al consesso più importante al mondo, la la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, per buttare, come si suol dire, la palla fuori, ha parlato di fusione nucleare. Fate pace con voi stessi, ma soprattutto siate chiari con gli italiani verso la direzione che il nostro Paese deve prendere sulla transizione energetica. In sostanza, per molteplici ed evidenti ragioni, il Governo italiano continua con ambiguità e colpi di scena a rallentare la transizione ecologica, che bolla strumentalmente come ideologica, non avendo argomenti, idee, coraggio e autonomia. Inoltre, il Governo distorce il dibattito sulla transizione ecologica e ostacola azioni rapide e concrete contro la crisi climatica. Sempre nel suo intervento a Baku, Meloni ha difeso un approccio di neutralità tecnologica, affermando che non esiste una soluzione unica alla transizione energetica. Tuttavia, queste posizioni distolgono l'attenzione dalle tecnologie già disponibili e più efficaci, per esempio, le rinnovabili. Il discorso della Presidente del Consiglio alla COP29 è emblematico in senso assolutamente negativo. Si è trattato di un discorso lontano dall'urgenza della crisi climatica, rivolto a tecnologie marginali e del tutto chiuso rispetto alla necessità di un rapido sviluppo delle energie rinnovabili. Proprio in quel contesto, la Presidente del Consiglio ha confermato come il proprio Governo si ponga malissimo verso la tutela dell'ambiente e del pianeta. Allo stesso tempo, quel discorso ha mostrato al mondo le resistenze, le tare e i paraocchi che in materia ambientale caratterizzano l'operato del Governo. Ecco perché non si capisce e non ci stupisce che ora discutiamo l'ennesimo

Ecco perché non ci sorprende l'ennesima riprova dell'improvvisazione dozzinale del Governo, che va avanti con decreti-legge concepiti in questo modo, all'ultimo momento, pieni di criticità e contraddizioni purtroppo insanabili, alla luce dei tempi e delle modalità di conversione. Hanno ragione i colleghi di maggioranza: il Governo ha totalmente svilito

veramente la responsabilità e il ruolo dei senatori sia di maggioranza sia di minoranza. Ecco è la novità di queste ore e di queste settimane: la divisione profonda all'interno della maggioranza, i cui colleghi a loro volta hanno dovuto tacere di fronte ai cambi immediati e repentini del Governo rispetto ai pareri sugli emendamenti. Tutto questo è inaccettabile per poter lavorare. Condivido l'appello che è stato fatto anche da qualche collega di maggioranza. Bisognerebbe iniziare a dare più autorevolezza e tornare alla centralità del Parlamento e al ruolo delle Commissioni. Ponendo la fiducia quindi il Governo giustifica se stesso e si legittima con il voto di una maggioranza critica, succube e rassegnata. Eppure anche stavolta avevamo avevamo cercato di contribuire con emendamenti puntuali a migliorare un testo di legge pieno di falle. Pensavamo al riuso delle acque per uso agricolo, pensavamo di ampliare la platea degli interventi e dei progetti sulle energie rinnovabili che potessero utilizzare potessero utilizzare la VIA semplificata; insomma, volevamo aiutare ad avviare un processo per modernizzare ed efficientare questo Paese. Ma avete detto di no. Semmai però, all'ultimo minuto, avete inserito un emendamento che introduce l'affidamento del servizio idrico a società *in house*. Leggo testualmente: «con partecipazione obbligatoria di capitali privati». Uno scandalo inaccettabile - inaccettabile! *(Applausi)* che si è bloccato grazie alla ferma opposizione in Commissione del Partito Democratico e di tutte le opposizioni, perché con un colpo di mano il centrodestra ha provato a cancellare la volontà che gli italiani hanno espresso in occasione del *referendum* sull'acqua pubblica.

a far entrare i privati. Se non è questa privatizzazione, collega Paroli, poi ci spiegate cos'è. *(Applausi)*. Dovevamo attenderci un'iniziativa del genere, perché è ormai chiaro che il Governo e la sua maggioranza perseguono interessi privati, calpestando la volontà e i diritti dei cittadini,

all'atto del ritiro di questo emendamento sono uscite delle notizie con affermazioni, da parte di membri del Governo e della maggioranza, secondo cui questo stesso emendamento sarà ripreso nella legge di bilancio o in altri provvedimenti. Noi vi diciamo con chiarezza: non riprovateci. *(Applausi)*. Faremo battaglia nelle Aule parlamentari e nel Paese e non vi consentiremo di far passare una norma tanto ingiusta e contraria ai principi fondamentali civili e democratici. Oltre a essere contrari a questo decreto, sia nel metodo che nel merito, siamo contrari all'indirizzo che questo Governo, privo di visione e di contatto con la realtà, ha dell'ambiente, della vita umana e del futuro delle nuove generazioni. Ogni volta, che si tratti di casa, circolazione stradale, giustizia, sanità, Regioni, bilanci, immigrati oppure ambiente, il Governo mostra arroganza, miopia, mancanza di rispetto per il Parlamento e per la democrazia, insensibilità, arretratezza, chiusura nel proprio sistema ideologico e soprattutto l'idea che gestire il potere non non comporti responsabilità nei confronti dei cittadini di oggi e di domani. Per tutti questi motivi, dichiaro il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. Il Governo ha perso un'altra occasione per lavorare a migliorare il futuro del nostro Paese. Signor Presidente, ho sentito dai banchi delle opposizioni arrivare a dire addirittura che con questo decreto-legge noi vorremmo fare un attacco alla transizione ecologica. In realtà questo decreto mette in evidenza in modo chiaro la determinazione di questo Governo a perseguire obiettivi fondamentali, quali la decarbonizzazione, l'implementazione delle energie rinnovabili, l'investimento nella sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente attraverso l'accelerazione delle bonifiche territoriali e l'adozione di misure necessarie per contrastare i fenomeni di siccità e prevenire il dissesto idrogeologico. Semplificare, velocizzare gli interventi e individuare delle priorità: sono queste le intenzioni contenute all'interno di questo decreto. Un decreto particolarmente atteso dagli enti locali e dagli operatori del settore, che si trovano spesso a fronteggiare una complessa burocrazia che talvolta mette a rischio la spesa di finanziamenti indispensabili, come quelli del PNRR. Infatti non è un caso - lo ricordava anche prima il senatore Paroli - che, durante le audizioni in Commissione, gli intervenuti abbiano sottolineato la validità e l'urgenza di questo provvedimento. Al contrario di quanto è stato detto dalle opposizioni in Commissione, è stato svolto un importante lavoro e consentitemi di ringraziare il presidente Fazzone, il vice ministro Gava, tutti i componenti della Commissione, i relatori Petrucci, Potenti e Rosso. L'Italia ha assunto a livello internazionale impegni rigorosi e ambiziosi di politica ambientale che intende raggiungere: questo è scritto nel decreto-legge in esame. Tra gli obiettivi strategici che si intende perseguire c'è l'autosufficienza energetica, un traguardo fondamentale per la nostra Nazione un obiettivo utile a garantire stabilità economica, ma anche ad evitare speculazioni sul costo dell'energia, spesso influenzato dalle instabilità geopolitiche a cui, purtroppo, negli ultimi anni ci siamo abituati. Investire nelle energie rinnovabili rappresenta lo strumento principale per realizzare la decarbonizzazione e, allo stesso tempo, assicurare la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'Italia. Vi era dunque la necessità di aggiornare il quadro normativo al fine di garantire una piena operatività agli attori della transizione ecologica. Era fondamentale snellire, razionalizzare e semplificare le procedure di valutazione ambientale, stabilendo criteri di priorità per la transizione nelle procedure di VIA e VAS in relazione a specifiche categorie di istanze legate alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile. Con il decreto priorità e accelerazioni degli investimenti per gli impianti ad idrogeno verde, generato da fonti rinnovabili, per i progetti fotovoltaici *offshore* e agrivoltaici, per il rifacimento e la ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari. Con questo decreto affrontiamo anche il tema delle bonifiche dei cosiddetti siti orfani, ovvero quei siti in cui non sono stati individuati i responsabili della contaminazione o dove non esistono soggetti che provvedano alle operazioni di bonifica. Sono le pubbliche amministrazioni a dover procedere alle bonifiche con proprie risorse per recuperare i terreni e per ridurre il loro impatto ambientale. Anche qui si sceglie di semplificare le procedure e ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo degli investimenti. Questo testo si occupa anche delle conseguenze della crisi climatica sul territorio, che provocano siccità e alluvione. Viene prevista una gestione più efficiente delle risorse idriche con interventi quali il ravvenamento dei corpi idrici sotterranei anche con acqua affinata. Lo ha ricordato anche il collega Paroli e lo voglio ancora una volta sottolineare: in questo decreto non c'è nessuna privatizzazione dell'acqua. Attenzione viene data al contrasto del dissesto idrogeologico, sempre con lo stesso approccio: agevolare i processi di attuazione degli interventi. Le statistiche ci dicono che la durata media per la realizzazione degli interventi in questo settore è di circa cinque anni: sono tempi troppo lunghi per prevenire e fronteggiare le calamità causate dai cambiamenti climatici. Sul dissesto idrogeologico vengono previsti i criteri per individuare le priorità di finanziamento, si inseriscono termini stringenti per l'assegnazione degli appalti e viene fatta una migliore allocazione delle economie derivanti dai piani straordinari di interventi. Viene infine avviato un censimento di tutti gli interventi a difesa del suolo per raccogliere e diffondere il quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto in Italia. Il decreto-legge che stiamo discutendo oggi rappresenta quindi un pilastro centrale per la politica del Governo Meloni e di Fratelli d'Italia, perché mira a raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica della nostra Nazione integrandoli con le richieste europee di sostenibilità, ma tenendo conto anche delle esigenze dei nostri sistemi produttivi e sociali. Sin dal suo insediamento, nel novembre 2022, il Governo Meloni ha posto l'ambiente e l'energia al centro della sua azione, come testimonia anche il Piano Mattei. Ricordo inoltre i provvedimenti adottati per mitigare l'aumento dei costi energetici, conseguenza del conflitto in Ucraina, e l'impegno nel soddisfare un crescente fabbisogno energetico. integrato energia e clima (PNIEC), trasmesso lo scorso luglio alla Commissione europea: un documento che ha ricevuto una valutazione positiva e che definisce chiaramente i nostri obiettivi per il 2030. A distanza di due anni, nonostante il contesto geopolitico si sia reso ancora più incerto di prima, ribadisco con fermezza che l'Italia continuerà a fare la propria parte nel processo di decarbonizzazione, attraverso un approccio più pragmatico e non ideologico ideologico al tema, attraverso una visione globale più realistica e più sostenibile, sia per l'ambiente che per le nostre aziende e per i nostri lavoratori. Un concetto, questo, ribadito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo recente intervento alla COP29 di Baku. Senatore Irto, le faccio notare che il presidente Meloni è stata uno dei pochi capi di Stato a partecipare alla COP29. Forse questo è qualcosa che le sfugge e che le è sfuggito nel suo intervento. Ma quale attacco, quindi, alla transizione ecologica? Bisogna bilanciare le esigenze di tutela ambientale con la salvaguardia della competitività delle nostre imprese. È questo l'approccio che deve essere usato anche per affrontare la crisi dell'*automotive* - di cui si è discusso ieri proprio qui in Senato - in Europa e in Italia. Su questo delicato tema, in Commissione è stato approvato anche un mio ordine del giorno, finalizzato al sostegno delle filiere dell'*automotive,* per garantire la continuità dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Bene ha fatto il ministro Urso, con il *non paper* per l'*automotive* presentato nell'ultimo Consiglio competitività a Bruxelles, a richiedere di riesaminare le modalità che porteranno allo stop dei motori endotermici nel 2035; una linea tenuta dall'Italia, che ha visto la condivisione di ben quindici Nazioni europee. Proprio ieri è stato ribadito dal ministro Urso alla Camera dei deputati che il Governo Meloni è pronto ad aumentare le dotazioni del fondo per l'*automotive* con risorse aggiuntive, ma servono prima chiari piani industriali, che restituiscano centralità agli stabilimenti italiani. Funziona così in Italia. Mentre c'è chi sceglie, nel nome della rivolta sociale, di indossare la casacca dell'opposizione, organizzando scioperi per contestare il Governo, c'è chi, fortunatamente, come il presidente Meloni, il suo Governo e la sua maggioranza, oltre a occuparsi di ambiente, lavora per tutelare lo sviluppo economico, i lavoratori, i loro salari, i loro diritti e per far crescere l'occupazione. Presidente, vista l'importanza di questo decreto-legge e per lo straordinario lavoro che il Governo Meloni sta portando avanti in Italia e in Europa, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla fiducia al Governo Meloni.

buona parte degli altri Gruppi di opposizione, ha depositato una mozione, che chiediamo venga calendarizzata al più presto. Mi auguro che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sempre molto celere nel trovare soluzioni che, purtroppo, a volte risultano rabberciate, come ci ha ricordato oggi il vice presidente del Gruppo Forza Italia, senatore Paroli, venga incontro alle esigenze delle opposizioni e possa aiutarci a discutere presto una mozione che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale Lo diciamo perché il ministro Calderoli ha annunciato di voler andare avanti nella stipula delle intese, indipendentemente dai tempi del Parlamento e dal recepimento dei rilievi della Corte costituzionale. Io sono convinto che le colleghe e i colleghi della maggioranza vogliano venire incontro alle richieste dell'opposizione, anche per rispetto del Parlamento. Signor Presidente, lo dico nel giorno della settantaquattresima fiducia: questa settimana ne avete chieste tre e presumibilmente, signori del Governo, otterrete anche questa. Io penso che con questo atteggiamento si stia sempre di più svuotando il Parlamento e delegittimando la nostra funzione. Per questa ragione, chiediamo con urgenza la calendarizzazione di questa mozione. Io mi auguro si possa discutere e votare insieme lo stop al ministro Calderoli della sottoscrizione, ma anche della proposta delle intese, fino a quando non saranno recepiti tutti i rilievi della Corte costituzionale. *(Applausi)*.

assieme a tante altre forze di opposizione. Ciò perché riteniamo che l'autonomia sia un tema serio, che vada seriamente affrontato nelle aule parlamentari, con un dibattito dibattito ampio in cui il Parlamento sia al centro e non al traino del Governo, che sa solo porre fiducie, anche su decreti in prima lettura, in un'Aula in cui l'ostruzionismo non esiste. esiste. Se questo è l'atteggiamento del Governo, io credo che si debba fare un fronte comune per evitare che si perseveri in questo atteggiamento. Abbiamo detto mille volte che i temi dell'autonomia, previsti dalla nostra Costituzione, vanno affrontati con un dibattito aperto, che voglia portare a compimento quegli spazi di sussidiarietà del territorio rispetto al Governo centrale, che sono previsti nella nostra Costituzione, ma che invece questo Governo, in particolare una forza politica di questo Governo, sta cercando di portare all'attenzione soltanto come una propria bandierina politica, senza dare risposte su questo al Paese. Pertanto, chiediamo con forza la calendarizzazione di questa mozione, ma soprattutto chiediamo la disponibilità del ministro Calderoli e del Governo ad iniziare un dibattito serio nel merito. *(Applausi)*.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

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*. *(La seduta, sospesa

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro dell'istruzione e del merito.

finestra") *(IV-C-RE)*. Signora Ministro, lei sa che la sua nomina in questo Governo per noi era stata una specie di luce, abbiamo ritenuto il fatto che un sincero garantista come lei, una persona i cui scritti e la cui opera per tanti anni aveva tenuto posizioni rigidamente garantiste, fosse un bene per il Paese e quindi, essendo noi anche all'opposizione, l'abbiamo sostenuta, tra l'altro votando alcuni provvedimenti da lei proposti, il che ci ha anche attirato qualche critica, diciamo la verità. Devo dirle, però, dopo due anni dal giorno in cui venne in Commissione dirci delle sue linee programmatiche (io ero lì), che il bilancio è molto, molto deludente. Lei è il rappresentante di un Governo che ha utilizzato il diritto penale in modo opposto a come lei lo ha sempre raccontato. Questo è un Governo schiettamente ruspante in termini di giustizialismo, che utilizza la norma penale come una sorta di panacea: ogniqualvolta c'è un problema nel Paese o un allarme sociale, in Commissione giustizia arrivate con una norma penale, con nuovi reati, spesso spesso tra l'altro scritti in decreti-legge, quindi in provvedimenti d'urgenza che non sono stati discussi, e per i quali non possiamo fare delle audizioni. Quei decreti-legge recanti norme penali, che quindi incidono sulla libertà dei cittadini, poi li emendate anche, perché sapete che vengono scritti male e quindi in corso di conversione siete anche costretti a modificarli, quindi abbiamo anche un caos nell'applicazione di queste norme penali,

Avete, con questa normativa in materia penale così ipertrofica, così insistita, che è quasi un manifesto, riempito le nostre carceri fino a farle esplodere: registriamo ormai 85 suicidi in un anno, una cosa, signor Ministro, che è insopportabile per la coscienza di un Paese civile. tutto questo avviene sotto la guida di una persona come lei che noi consideravamo e consideriamo un sincero garantista, uno che diceva che avrebbe ridotto i magistrati fuori ruolo (e i magistrati fuori ruolo sono tutti lì), che avrebbe fatto funzionare le misure alternative (e i braccialetti elettronici non funzionano). Insomma, signor Ministro, lei ha in mano un Ministero della giustizia che è tutto il contrario di quello che lei rappresenta: mi racconta come è andata e cosa intende fare per cambiare rotta?

un grande politico inglese diceva che ci sono delle persone che abbandonano le proprie idee per amore del partito e delle persone che abbandonano il partito per amore delle proprie idee.

È vero che abbiamo aumentato il numero dei reati, ma questo dipende dal fatto che vi sono dei vuoti di tutela che si presentano anche, per esempio, a causa dell'evoluzione tecnologica. I grandi reati che si commettevano una volta, per esempio le rapine a mano armata in banca, stanno scemando perché la banca non ha più il *cash* al proprio interno, essendo il denaro dematerializzato, mentre aumentano le frodi informatiche e ora con l'intelligenza artificiale aumenteranno altre forme di delinquenza. Questi vuoti normativi vanno colmati. Faccio solo un esempio per per quanto riguarda il rapporto tra novità normative e sovraffollamento delle carceri. Il primo provvedimento che noi abbiamo adottato è stato quello criticatissimo sui *rave party.* Sapete quante persone sono finite in prigione per i *rave party*? Nessuna. persone probabilmente abbiamo evitato che entrassero in prigione con l'adozione della norma sui *rave party*? Statisticamente abbastanza, se non come condanne definitive, quantomeno come arresti. arresti. Abbiamo anche deflazionato il codice penale sostanziale: secondo me, l'abolizione del reato di abuso di atti di ufficio vale da solo l'introduzione di una ventina di nuovi piccoli reati, che sono stati degli assestamenti dovuti soprattutto ai vuoti di tutela determinati dall'avanzare tecnologico.

auspichiamo, direi che siamo certi che avremo la doppia lettura entro la fine della primavera o all'inizio dell'estate. Quella sul braccialetto elettronico è una questione estremamente complessa e tecnica. Noi abbiamo introdotto la norma che adesso garantisce l'operatività del braccialetto elettronico caso per caso, dando al giudice e alla polizia gli strumenti per valutare, nel momento del *warning,* dell'allarme, del pericolo, la possibilità di limitare il rischio di avvicinamento tra persone a rischio. intervenire in replica il senatore Scalfarotto,

è che in uno Stato di diritto più sono i reati, meno sono gli spazi di libertà e questo, signor Ministro, non le assomiglia, però assomiglia molto a una persona che collabora con lei, cioè il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che ha un'idea della giustizia molto diversa dalla sua. È quello che, davanti alla tragedia delle carceri, dice che lui non si inchina alla Mecca dei detenuti, per dire che non va a verificare lo stato delle carceri; è quello che al giuramento della Polizia penitenziaria fa fare agli

- non respirano. Questa legislazione così pesante in materia penale assomiglia molto al sottosegretario Delmastro Delle Vedove e stupisce il fatto, signor Ministro, che lei non si faccia valere, che non faccia trasparire in filigrana la sua visione visione della giustizia. Io credo che questo non faccia onore alla sua storia, alle cose che ha fatto e alle cose che ha scritto. Penso - e mi perdoni se glielo dico che forse, dato che alla fine la responsabilità di tutto quello che viene deciso è sua, una riflessione se non valga la pena di staccarsi da quella responsabilità politica io la farei.

dalla nostra Costituzione, è una norma di mero principio, del tutto scollegata dalla realtà fattuale. Pertanto, è assodato che la pubblica accusa seleziona le notizie di reato secondo alcuni criteri che noi ci auguriamo essere i più obiettivi possibili. Proprio per garantire ordine e trasparenza si sono adottati nel tempo i cosiddetti criteri di priorità fissati dalle tabelle delle singole procure. iniziò per primo il procuratore Maddalena di Torino (con la famosa circolare Maddalena) e poi sono seguite iniziative di diverse procure. Ognuna si è fatta la sua circolare con i propri criteri di priorità. Proprio per garantire

Signor Presidente, senatore Zanettin, come lei ha opportunamente ricordato, ci troviamo di fronte a una norma costituzionale primaria

Lei ha giustamente ricordato le iniziative, prima, delle procure della Repubblica e, poi, del Consiglio superiore della magistratura che, potrei aggiungere, non sono e non erano vincolanti, proprio perché ogni magistrato, ossequioso al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale scritto in Costituzione, si riteneva - secondo me giustamente - in diritto di procedere secondo le sue intenzioni, anche se poi di fatto, come sappiamo (io condivido le sue osservazioni), l'azione penale era diventata discrezionale o addirittura arbitraria. Dopo la cosiddetta legge Cartabia, il Parlamento deve dare questi indirizzi generali, ai quali - poi - le procure dovranno in un certo senso uniformarsi, quantomeno sotto gli aspetti organizzativi, fermo restando che, rimanendo l'obbligatorietà dell'azione penale, il loro perimetro di intervento sarà limitato.

Poi, se tutto è priorità, niente diventa più priorità, quindi è una notevole responsabilità, vorrei dire parlamentare, alla quale certamente il Governo e il Ministero si associano, proprio come studio e contributo per arrivare a una soluzione soddisfacente, che lo sia anche per le procure, perché se poi le procure della Repubblica, anche in base a questa legge e a questo indirizzo, si discostano, invocando la fonte primaria della Costituzione, che è l'obbligatorietà dell'azione penale, la questione si complica ancora. Quindi, in conclusione, il Governo e il Parlamento, compresa maggioranza e opposizione, è bene che lavorino insieme per trovare un indirizzo unitario, condiviso possibilmente anche con il Consiglio superiore della magistratura.

della sua risposta. Mi pare che condividiamo in tutto e per tutto quello che deve essere il percorso da svolgere, tant'è che credo che questo debba essere segnalato. Ho sempre detto, anche nel corso del dibattito in Commissione giustizia, che l'iniziativa del singolo parlamentare, quale posso essere io, fosse solo di stimolo, ma il vero impulso dovesse arrivare dal Governo, perché solo il Governo è in grado di avere tutti i dati relativi al territorio nazionale, per fare delle scelte, che

dell'occasione, di dichiarare che sono rimasto molto sorpreso dalle reazioni di molta magistratura a seguito delle anticipazioni del vice ministro Sisto, che ha gridato allo scandalo, perché si vuole lavorare su questa materia. Probabilmente questi pur illustri magistrati che hanno rilasciato le loro interviste non avevano capito che la norma era già contenuta nella legge Cartabia, una legge che - ripeto - abbiamo votato praticamente tutti all'interno del Parlamento dopo un percorso di condivisione e di studio molto

lunedì 25 novembre 2024 è stata celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni unite tramite la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999. Nell'ultimo decennio, il fenomeno della violenza sulle donne ha assunto un carattere di allarme sociale e messo in evidenza un vuoto culturale che deve essere sanato attraverso una rinnovata e profonda educazione civica, specialmente rivolta alle nuove generazioni. Questo percorso per raggiungere i suoi obiettivi avrà bisogno di essere affrontato nel lungo periodo. È per questo che il legislatore al contempo ha avviato, attraverso importanti modifiche normative, strategie atte a contrastare la crescita esponenziale dei femminicidi e la violenza contro le donne. Negli ultimi anni tutte le forze politiche, quando hanno assunto responsabilità di Governo, tanto hanno fatto: basti pensare alle norme che hanno inasprito le pene contro lo *stalking*, fino all'introduzione del cosiddetto codice rosso. Con quest'ultimo il legislatore ha infatti introdotto norme e pene più severe contro la violenza sulle donne. Grazie a ciò è maturata una consapevolezza maggiore da parte delle donne e un rinnovato sentimento di fiducia nelle istituzioni. Queste modifiche normative hanno teso ad accorciare i tempi di intervento da parte delle autorità, rassicurando le donne e offrendo loro protezione nel momento in cui decidono di denunciare. In particolare, secondo quanto previsto dal cosiddetto codice rosso, oggi l'autorità giudiziaria deve ascoltare la vittima entro tre giorni dall'avvio del procedimento. Il magistrato può valutare subito la gravità della situazione dalla viva voce di chi denuncia. Nel settembre 2023, il legislatore ha fatto un importante ulteriore passo in avanti andando a rafforzare il codice rosso, prevedendo che, se una donna che denuncia non viene ascoltata nei tre giorni stabiliti, il procuratore capo può assegnare il fascicolo ad un altro pubblico ministero o occuparsi direttamente del caso. Grazie che vivono una concreta situazione di pericolo e allo stesso tempo mettere in campo attività di sensibilizzazione ed educazione, affinché questi atti delittuosi diventino finalmente un brutto ricordo, si chiede di sapere quali ulteriori attività di propria competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno mettere in atto al fine di rendere maggiormente operative le modifiche normative varate in questi anni.

questa volta, invece di censurare l'opera del Governo e del Parlamento per una iperproduzione normativa penale, si prende invece atto che non solo per un vuoto di tutela, ma per una maggiore sensibilità verso questa problematica così lacerante, abbiamo effettivamente inasprito le pene e introdotto non solo nuovi reati, ma concepito una migliore procedura, quella che lei ha appena enunciato e sulla quale non mi soffermo, relativa al Codice rosso e ai doveri del procuratore della Repubblica. Credo che per quanto riguarda il diritto sostanziale,

anche per una ragione che, tra l'altro, condividiamo perfettamente con i colleghi, in particolare con il collega Valditara e con la collega Roccella; questo fenomeno, ripeto, lacerante e doloroso, quasi sacrilego, vorrei dire, del femminicidio e della violenza contro i soggetti deboli, donne in particolare, ma anche i bambini, vada, sì, represso, perché lo Stato deve affermare la sua autorevolezza e anche agire in senso deterrente attraverso delle pene che siano non dico esemplari, ma rigorose, proporzionate e certe, ma soprattutto deve agire in via preventiva attraverso l'educazione. È un'educazione che deve cominciare addirittura, prima ancora che dalle scuole, dalle famiglie, perché è lì che si forma il *software* del bambino che poi, sviluppandosi, diventerà rispettoso dei diritti altrui, cercando di vedere

i commissariati delle Forze di polizia di Italia, in modo da avere un quadro praticamente in tempo reale di tutto ciò che accade e che viene gestito sia nell'ambito della Polizia e delle indagini preliminari sia nell'ambito giudiziario. Abbiamo fatto anche qualcosa di più di più accessibile, stampando migliaia e migliaia di piccole pubblicazioni che contengono i segnali di allarme che devono che devono indurre la donna a rivolgersi al più vicino posto di polizia o altro per ottenere protezione, anche attraverso un'attività informativa che, per esempio, a molti è ignota. Mi riferisco ad esempio al fatto che le donne hanno diritto a un'assistenza legale che, in questi casi, è non tutti conoscono. Per quanto riguarda il braccialetto elettronico, abbiamo introdotto una norma, ma soprattutto stiamo lavorando di concerto con la Polizia, per rendere realmente efficace questo sistema che ha effettivamente mostrato alcune difficoltà, soprattutto vista vista la distanza ravvicinata tra potenziale vittima e potenziale aggressore che oggi è colmabile in pochi minuti, mentre il braccialetto elettronico manda un *warning*, che molto spesso è insufficiente.

restituirà queste splendide donne; ma chi minaccia, maltratta o peggio ancora uccide una donna va perseguito senza indulgenza. Ministro, vi è un altro tema da affrontare per evitare che al dolore si aggiunga ulteriore dolore, se non una beffa: il Gruppo Lega, ha presentato una proposta di legge che vuole evitare l'inquinamento delle prove in alcuni processi. Ad oggi, a legislazione vigente, un soggetto iscritto nelle notizie di reato per un femminicidio può scegliere di cremare il corpo della vittima. In questo modo, però, può disperdere delle prove essenziali, perché a volte sul cadavere si possono fare delle analisi. Questo può accadere perché quel soggetto è il coniuge un parente, e questo è inaccettabile. Approfitto della presenza del ministro Valditara per complimentarmi con lui per l'incontro con Gino Cecchettin, che ha portato alla definizione di possibili interventi tra la Fondazione Cecchettin e il Ministero, per individuare azioni comuni volte a combattere non solo il femminicidio, ma ogni forma di violenza. Questa sinergia rappresenta un ottimo strumento per concretizzare la cultura del rispetto e dell'educazione, partendo dalla scuola, ma - come diceva il Ministro - anche dalla famiglia. Rispetto verso tutte le donne. Le donne hanno lottato anni per i propri diritti e nessuna cultura o religione le può considerare esseri inferiori. Tali battaglie non devono essere strumentalizzate e non devono essere di destra o di sinistra, ma sinergiche, perché questi orribili reati non accadano più.

Signor Presidente, signor Ministro, premesso che dall'agenda del G7 giustizia svoltosi a Venezia nel maggio scorso è nato il Venice justice group, per rafforzare e coordinare le iniziative degli Stati membri del G7 rispetto alle nuove sfide globali nel campo della giustizia e della difesa dello Stato di diritto, il 14 novembre scorso, nella sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si è tenuta la prima riunione del G7-Venice justice group, a cui ha preso parte anche una delegazione dell'Unione europea. Il gruppo di lavoro ha posto al centro del dibattito l'impatto dell'intelligenza artificiale nel campo della giustizia, condividendo all'unanimità l'obiettivo di promuovere una giustizia sempre più digitale, inclusiva e trasparente, che metta la tutela dei diritti al centro di ogni innovazione tecnologica. Considerato che il 23 ottobre 2024 si è reso operativo, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale, uno strumento fondamentale per garantire che l'innovazione tecnologica sia al servizio della giustizia e dei cittadini, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali e nelle attività strumentali della giurisdizione, al fine di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l'efficienza e la qualità del sistema giuridico al servizio dei cittadini e, al contempo, garantire la centralità dell'uomo e della sua creatività. PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, onorevole Nordio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata,

in realtà portò la più grande rivoluzione religiosa della storia del cristianesimo, perché con i caratteri mobili di Gutenberg la Bibbia fu stampata in migliaia di copie ed entrò nelle case dei tedeschi, che incominciarono a leggere i testi sacri senza l'intermediazione della Chiesa e quindi passarono direttamente dalla parte di Lutero, eliminando la devozione alla Chiesa cattolica. È un esempio che, secondo me, me, dovrebbe illuminarci sul fatto che l'intelligenza artificiale in questo momento è un elemento misterioso, che noi conosciamo solo in parte, di cui dobbiamo tener presente il grande pericolo, ma anche la grande opportunità. L'intelligenza artificiale applicata alla giustizia non potrà mai sostituire il cervello umano, questo è ovvio. Essa potrà infatti aiutare il giudice nell'elaborazione del diritto e nella

ma non potrà mai raggiungere, per esempio, la ricostruzione del fatto e tantomeno l'elemento psicologico che sta alla base del fatto, perché un reato può essere commesso con colpa, con dolo, con premeditazione, con preterintenzione. In tutto questo l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il giudice e noi stiamo operando in questo senso, tant'è vero che le prime normative che abbiamo elaborato sono indirizzate nell'unica funzione di agevolare il giudice nella sua ricerca organizzativa e giurisprudenziale, ma senza entrare nel merito. Vorrei però aggiungere, in conclusione, che - dobbiamo evitare di trovarci impreparati di fronte a questo nuovo strumento tecnologico, trasformandolo invece in opportunità. Quello che dobbiamo fare, secondo me, è lavorare di fantasia, come avrebbe dovuto lavorare di fantasia Gutenberg quando fece i caratteri mobili. Il vero pericolo, infatti, non è tanto nella captazione dei dati, che già sta avvenendo, ma sarà nella manipolazione dei dati. L'intelligenza artificiale sarà in grado di manipolare, non in modo virtuale ma reale, quello che è un mondo che oggi può essere manipolato in modo grossolano. La fotocomposizione, il fotomontaggio è sempre esistito; oggi però si può fare in un nanosecondo usando le persone nella loro realità. Ecco, dobbiamo intervenire preventivamente lavorando di fantasia, immaginando questi tipi di reati. Infatti, essendo la legge penale - come sapete - non retroattiva, non possiamo trovarci impreparati nel momento in cui l'intelligenza artificiale si manifestasse attraverso forme criminose che non siano coperte da una normativa repressiva. Ecco, questo è il nostro compito e su questo stiamo studiando. Abbiamo

che vuol dire oggi l'intelligenza artificiale. La politica, da una parte, quindi il legislatore e anche il Governo si devono preoccupare di quelli che possono essere gli eccessi dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto di come mantenere sempre l'uomo al governo dell'intelligenza artificiale, non solo sfruttandola al meglio per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, come ha accennato lei, ma anche nel saper combattere l'intelligenza artificiale come fonte di reato. Anche su questo aspetto dobbiamo essere molto attenti, perché sappiamo bene, come il caso del lei ha citato, che ora siamo già ai filmati con voci di altri che mettono in bocca alle persone parole non dette, cose non fatte e fatti non avvenuti. C'è quindi un aspetto globale ed una ricerca globale di quello che dobbiamo fare, da una parte il legislatore e dall'altra parte il Governo, per far sì che l'uomo rimanga sempre al centro e l'intelligenza artificiale non abbia mai la supremazia sull'intelligenza e soprattutto sulle emozioni dell'uomo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, signor Ministro, l'Italia sta investendo da anni ingenti somme di denaro e risorse nell'acquisto dei caccia F-35 di produzione statunitense, un aereo da combattimento che ha già comportato un enorme impiego finanziario per il nostro Paese. Parallelamente, è stato recentemente avviato il programma Global combat air programme (GCAP), una collaborazione internazionale con il Regno Unito e il Giappone per lo sviluppo di un nuovo caccia bombardiere di sesta generazione che richiederà ulteriori e significativi investimenti. È emerso inoltre che anche l'Arabia Saudita sarebbe interessata e potrebbe entrare a breve nel progetto, sollevando così interrogativi sulle implicazioni geopolitiche e sulle eventuali ripercussioni economiche. Sul programma F-35, che noi abbiamo sempre considerato un pessimo investimento, personalità di rilievo internazionale come Elon Musk, un vostro sostenitore, hanno espresso dubbi sulla reale efficacia. In particolare, Musk ha recentemente dichiarato che l'F-35 non sarebbe in grado di competere con sistemi di combattimento aereo basati su droni e intelligenza artificiale, dichiarando senza mezzi termini che non ci investirebbe più nemmeno un dollaro. Nel frattempo, Francia, Germania e Spagna stanno sviluppando un loro programma aereo, il Future Combat air system (FCAS/SCAF), che coinvolgerà a breve anche il Belgio e che potrebbe drenare significativi fondi europei per la difesa europea verso questa iniziativa, limitando così le risorse disponibili attualmente per altri programmi in essere a livello continentale, tra cui anche quelli che già coinvolgono l'Italia. In Commissione, qualche giorno fa, il Capo di stato maggiore della Difesa ha espresso preoccupazione riguardo alle limitate risorse disponibili: mancanza di personale civile e militare e mancanza di fondi per le spese di esercizio e/o per la formazione dei nostri militari, elementi fondamentali per garantire l'efficienza e la prontezza operativa delle Forze armate. Le chiedo quindi, signor Ministro, se non ritiene opportuno riconsiderare l'investimento previsto di 7 miliardi per l'acquisto di ulteriori cacciabombardieri F-35, valutando magari delle alternative che possano garantire comunque la sicurezza nazionale senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato e come si concilia l'impegno del costoso programma GCAP, soprattutto considerando l'eventuale ingresso dell'Arabia Saudita e ciò che ne consegue, con le attuali limitazioni di bilancio che penalizzano le spese di esercizio e la formazione del personale militare. In ultimo, le chiedo quali misure intende adottare per assicurare una gestione più efficiente delle risorse destinate alla difesa, considerando anche l'impatto negativo che il programma di Francia e Germania potrebbe avere sui fondi europei disponibili per l'Italia.

F-35. La scelta di aderire al programma relativo a un veicolo di quinta generazione, come lei sa perfettamente, senatore, è stata presa quasi trent'anni fa ed è stata sempre avallata da tutti i Governi che in questi trent'anni si sono succeduti, compreso il Conte I e il Conte II, ma si è dimostrata nei fatti finora corretta. Nel mondo sono stati complessivamente consegnati oltre 1.000 di questi aerei, sono stati addestrati oltre 2.600 piloti e sono state effettuate oltre un milione di ore di volo complessive. Sotto il profilo qualitativo, oltre al vantaggio operativo e al potenziamento della capacità di difesa e deterrenza, il programma F-35 - lei sa benissimo - ha accelerato l'acquisizione di competenze tecnologiche con ricadute positive, ma in campo duale, non soltanto in campo specificamente militare, sia sul lungo termine, sia in tutti i settori della difesa e in prospettiva anche in termini occupazionali sull'industria civile. Il polo tecnologico trivalente regionale europeo di Cameri è ormai da tempo un esempio concreto e anche unico nel mondo che quasi tutti i Paesi europei invidiano delle ricadute del programma F-35 e uno dei tre soli stabilimenti nel mondo in grado di assemblare un aereo di questo tipo e l'unico presente in Europa. Ora a Cameri vengono assemblati i velivoli destinati a Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, questo per spiegare che quell'investimento ha avuto ricadute ulteriori che vanno al di là della valenza per la difesa di questo aereo.

che io però condivido, perché alla fine è uno strumento di deterrenza unico al mondo - ma ha garantito anche una ricaduta sociale significativa. Il programma GCAP è molto più recente. Nasce con una firma del ministro Elisabetta Trenta durante il Governo Conte I,

i Paesi sia importante dal punto di vista sia tecnologico, sia economico e che il fatto che altri Paesi vogliano associarsi sia indice della fiducia che questo programma sta ispirando nel mondo. nel mondo. Il Parlamento ha approvato il trattato; è in fase d'avvio la *joint venture* industriale. La nostra partecipazione ci porterà a un accesso a un'*élite* tecnologica di assoluta eccellenza nel mondo. Può essere un punto di svolta nel campo aerospaziale che, come lei sa, va in quella linea che ha indicato Elon Musk, perché va in una linea di sesta generazione che possa superare anche l'elemento umano nel volo, che è la sintesi del ragionamento di Musk di cui lei ha parlato. Quindi è un salto con cui si guarda in avanti; non dovrebbe esserci una competenza sui fondi europei del progetto franco-tedesco-spagnolo, che però, a quanto ci è dato di sapere, non ha prospettive di crescita pari a quelle del GCAP, anche perché tutti questi programmi poggiano quasi esclusivamente su risorse delle Nazioni che ne fanno parte. Per quanto riguarda una gestione più efficiente delle risorse destinate alla difesa, io sposo quello che ha detto il senatore Marton e sposo le preoccupazioni del capo di Stato maggiore della difesa. Probabilmente non ci si è resi conto della gravità nei tempi in cui viviamo e della necessità di aumentare gli investimenti della difesa, nell'approntamento delle truppe,

tutti i Governi si sono impegnati ad arrivare al 2 per cento entro il 2028. A questo punto, non posso che manifestare una mia preoccupazione per la possibilità di arrivare a quel risultato, se non cambieremo le regole europee. Mi ostino a dirlo da due anni; finora non è stato colto da nessuno, ma c'è un limite che ci verrà

Mi pare di aver capito che si continuerà a spendere soldi per gli F35; è evidente che continueremo a investire sette miliardi su questo aereo. Il Ministro non ha risposto, o meglio ha risposto tentennando sul fatto che il GCAP possa essere in concorrenza con il il sistema aereo francese, tedesco e spagnolo e che questo possa drenare risorse. È evidente che lo farà, signor Ministro: noi ci troveremo a far concorrere prodotti europei con un prodotto extraeuropeo e immagino che tutta l'Europa andrà dietro a Francia e Germania. È una mia preoccupazione, quindi la invito a vigilare affinché ciò non avvenga. Signor Ministro, andiamo in un programma extraeuropeo, alla faccia della difesa comune che tanto abbiamo propagandato. È evidente che stiamo abbandonando la difesa comune con un programma extraeuropeo. Continueremo quindi a spendere montagne di denaro pubblico e lasciamo i nostri soldati con

Signora Presidente, signor Ministro, illustro un quesito decisivo e a nostro parere fondamentale per il benessere e il funzionamento della scuola pubblica italiana, All'articolo 110 del disegno di legge di bilancio si stabilisce, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia, con corrispondente riduzione del personale docente previsto a legislazione vigente.

oltre 88 milioni di euro per il 2025 e ben 267 milioni di euro dal 2026, che incideranno negativamente sul sistema scolastico. Come la stessa Corte dei conti in sede di audizione ha osservato, sono minori risorse su cui non è avvenuta una valutazione dei loro effetti sulla formazione delle classi e sul corretto avvio delle lezioni, manovra non sono per nulla specificati i criteri che dovrebbero gestire successive rimodulazioni. Invece è sempre più ribadita la necessità di invarianza finanziaria. D'altra parte, le risorse destinate al rinnovo del contratto del personale della scuola appaiono insufficienti e inadeguate, senza che siano stati stanziati i fondi per innalzarne le retribuzioni e garantirne definizione e progressioni di carriera per andare incontro agli *standard* europei. Allo stesso modo, vi è assoluta mancanza di certezza sull'assunzione e stabilizzazione dei docenti di sostegno e non ci sono nemmeno risorse previste per il diritto allo studio, libri e mobilità, né per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Solo tagli anche in questo ambito. Considerato che questi problemi sono dentro un disegno più ampio che sembra rivolto a sottrarre centralità all'istruzione pubblica (che, forse va ricordato, non è un conto corrente da cui fare cassa per sanare il Paese, impoverendola e rendendola più fragile nell'edificare e cementare cittadinanza responsabile), chiediamo, Ministro, quali iniziative intende intraprendere per sottrarre il sistema scolastico pubblico agli effetti della riduzione del 25 per cento del *turnover* nella pubblica amministrazione e far fronte al prospettato taglio di circa 8.000 unità di personale scolastico tra organico dell'autonomia e personale ATA; assicurare nuove assunzioni e stabilizzazioni dei docenti di sostegno che siano adeguate alla crescente richiesta di inclusione e formazione degli alunni con disabilità; sostenere e promuovere il sistema di istruzione pubblica, imprescindibile per garantire una democrazia equa, giusta, solidale e plurale, come sancito dalla nostra Costituzione. PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione e del merito, professor Valditara, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, gentili senatori, voglio subito rimarcare l'operato del Governo che, anche in questa legge di bilancio, ha fatto sì che ci fosse una crescita complessiva degli investimenti per il sistema scolastico. Come si legge nel *dossier* redatto dalla Camera dei deputati (non sono dunque congetture di parte, ma è un atto neutro), rispetto al 2024 il disegno di legge di bilancio 2025-2027 evidenzia per il Ministero dell'istruzione e del merito un notevole incremento nel 2025, un notevole incremento nel 2025, in termini assoluti pari a 4,6 miliardi di euro (più 8,9 per cento). Inoltre, con riferimento ai soli interventi legislativi, la manovra finanziaria per il 2025 determina complessivamente un incremento delle spese finali di 216,6 milioni di euro. A ciò aggiungo che, per il rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del pubblico impiego, quindi anche del personale scolastico che ne costituisce una componente molto importante, abbiamo ottenuto, come da me richiesto, un ulteriore aggiustamento, sino ad arrivare al 6 per di aumento. Peraltro, con il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40.000 euro lordi, tutto il personale della scuola godrà in via definitiva di tale beneficio, che ne accrescerà il potere di acquisto. Ancora, per la prima volta nella storia della contrattazione pubblica, sono già state stanziate risorse per la successiva tornata contrattuale 2025-2027,

Con queste risorse si riconosceranno incrementi retributivi al personale della scuola pari al 5,4 per cento a regime superiore all'inflazione programmata e con le erogazioni dei primi anticipi già nel 2025. nel disegno di legge di bilancio è stato istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con uno stanziamento di 122 milioni per il 2025, 189 milioni per il 2026 e 75 milioni di euro a partire dal 2027. Si tratta di risorse nuove, che è mia ferma intenzione utilizzare, fra l'altro, per l'avvio di un piano importante di stabilizzazione dei docenti di sostegno, che nel nostro auspicio consentirà di assumere un numero di insegnanti addirittura superiore rispetto ai tagli di organico attualmente previsti. Quanto fin qui da me illustrato dimostra un saldo positivo tra i nuovi investimenti e il contributo che, al pari di tutti i Ministeri, anche il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito per consentire le misure di una legge di bilancio equilibrata ed attenta in particolare alle esigenze dei ceti meno abbienti e, come detto, del pubblico impiego e del personale della scuola in particolare. Ciò premesso, in ogni caso stiamo verificando anche la possibilità di rimodulare i tagli di organico attualmente presenti, valutandone le effettive conseguenze in relazione al fenomeno del decremento demografico e della riduzione della popolazione studentesca. Questi tagli in ogni caso, è bene dirlo è bene dirlo anche con molta chiarezza, a differenza di quanto riferito nell'interrogazione, sono inferiori in termini assoluti a quelli, pari a 9.550 unità, effettuati dal ministro Bianchi del Partito Democratico. *(PD-IDP)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, però noi siamo molto preoccupati e non siamo soddisfatti delle parole che abbiamo qui sentito. Sembra che abbiamo letto tabelle diverse e conti diversi. Intanto, c'è un taglio del personale - ed è questo che noi volevamo sottolineare - ed erano anni che non c'era un taglio così preciso del personale dell'organico, in particolare, signor Ministro, degli ATA. Lei si ricorderà che sugli ATA i tagli del 2008 ebbero un fortissimo impatto e colpirono in modo durissimo: furono 45.000 quelli tagliati e da allora la scuola ha un problema in questo campo. A ciò si aggiunge che, essendoci stato il dimensionamento della rete scolastica, anche questo deciso in particolare da una vostra legge di bilancio del 2023, noi abbiamo una situazione di grande sofferenza sul personale, che è un pilastro è un pilastro fondamentale per il funzionamento delle scuole: c'è grande sofferenza proprio sulle succursali, che non sono più sedi centrali, e sul modo in cui la scuola si è riorganizzata. I soldi per i contratti in realtà non bastano: stiamo parlando di un tasso di inflazione reale che ormai è considerato al 18 per cento, quindi le cifre che lei ha dato non sono sufficienti. Rimane un grande dubbio: lei sta pensando di lei sta pensando di rimodulare e andremo a vedere come; ad oggi quello che c'è è il taglio e quello che c'è è un fondo che non si capisce come potrà garantire un piano di assunzione straordinario degli insegnanti di sostegno, la cui richiesta, a fronte di una diminuzione della platea di ragazzi e ragazze, è aumentata del 6,4 per cento. Forse la denatalità poteva essere l'occasione di ripensare il sistema, di evitare le "classi pollaio" e dare una maggiore offerta formativa di qualità. Invece noi la stiamo usando per tagliare e per diminuire l'offerta formativa. Le voglio anche ricordare che, se c'è stato un piano di assunzione, quello è stato fatto nel 2022: 25.000 insegnanti di sostegno, dei quali voi avete anche scelto, nell'ultimo decreto, di diminuire la qualità della formazione, il che significa anche diminuire la qualità dell'inclusione, all'istituto Indire la possibilità di corsi fatti di soli 30 crediti formativi universitari. Tutto questo ci fa dire che noi vigileremo, perché ci piacerebbe essere smentiti, ma quello che leggiamo nel disegno di legge di bilancio, purtroppo, è una secca diminuzione della capacità della scuola di sostenere il diritto allo studio, che è il diritto al futuro dei ragazzi e delle ragazze di questo Paese.

Signora Presidente, mi consenta, in chiusura della seduta di oggi, di svolgere un breve intervento raccomandando al nostro Governo la necessità di tutelare le comunità cristiane in Siria. signor Presidente, noi dimentichiamo che la Siria è un'autentica culla del cristianesimo. Pensiamo solo alla figura di San Paolo, che in realtà era Paolo di Tarso, o di San Simeone Stilita, un eremita ed asceta che passò la sua vita seduto sopra una colonna in una cittadina vicina ad Aleppo. Ormai da anni la comunità cristiana siriana è costretta a una drammatica diaspora. Il colpo di grazia rischia di assestarlo la recente offensiva dei ribelli sunniti provenienti da Nord, dalla sacca di Idlib. Per fortuna, finora questi hanno evitato violenze contro i cristiani, ma le preoccupazioni persistono. Poco fa le agenzie hanno battuto anche la notizia che sarebbe caduta, dopo Aleppo, anche la città di Hama, importante sulla strada di Damasco, che è stata abbandonata dalle forze del Governo siriano. Abbiamo ascoltato, Presidente, in questi giorni da Damasco le parole del cardinal Zenari, veneto, come il sottoscritto, nativo di Villafranca, in provincia di Verona, nunzio apostolico in Siria, una figura assolutamente straordinaria, non a caso creata cardinale da Papa Francesco, e che da molti anni si preoccupa della tutela delle comunità cristiane, senza averle mai abbandonate, in un territorio così difficile. Rivolgiamo anche un pensiero preoccupato ai frati francescani di Aleppo, il cui convento è stato bombardato pochi giorni fa. Per fortuna non ci sono state vittime, ma è stato bombardato e ha creato sicuramente grande sconcerto.

Una giornata che deve servire a rammentarci che cos'è il suolo e come sia direttamente collegato alla nostra quotidianità. Il suolo è una risorsa finita e non rinnovabile, necessaria per la nostra esistenza. Un ecosistema complesso, ricco di biodiversità, una sorta di spugna che incamera carbonio dall'atmosfera, quindi uno dei principali alleati nella mitigazione del cambiamento climatico. Il suolo ci regala gli alimenti sulle nostre tavole e quindi ci sfama con il 95 per cento del nostro cibo, ci fornisce acqua pulita e quindi ci disseta. Tra l'altro, per coincidenza, oggi in Aula si è parlato del provvedimento che riguardava anche la difesa del suolo, ma, ahimè, nulla è stato preso in considerazione a proposito della difesa di questo patrimonio comune e in via di estinzione. Alla parola suolo, infatti, dobbiamo inevitabilmente aggiungere la definizione del suo degrado, ossia il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo; più suolo consumiamo, meno servizi ecosistemici potranno Ecco perché la Comunità europea si è data l'ambizioso obiettivo di raggiungere un consumo di suolo netto pari allo zero entro il 2050 per tutti i Paesi membri. In Italia oggi abbiamo però davvero poco da festeggiare perché pochi giorni fa sono stati presentati da ISPRA i nuovi dati sul consumo in Italia, che continua a trasformare il nostro territorio con velocità elevate. Nell'ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 72,5 chilometri quadrati, ovvero, in media, circa 20 ettari al giorno, al ritmo di 2,3 metri quadrati ad ogni secondo; quindi 20 ettari al giorno in meno di servizi per tutti noi che si vanno a sommare a quelli sottratti negli anni precedenti. Sì, perché il consumo di suolo non si è mai fermato. Per raggiungere l'obiettivo del 2050 dobbiamo fare in fretta a cambiare il senso di marcia; non possiamo più consumare, ma dobbiamo restituire suolo. In Italia non c'è ancora una legge che tuteli la nostra risorsa. Ora più che mai diventa urgente una legge che

La seduta è tolta